recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE

Presidente stimatissimo, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il disegno di legge n. 2825, già approvato dalla Camera dei deputati il 14 luglio scorso, reca la conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89. Questo decreto, composto di sei articoli, dispone il completamento dell'attuazione della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini comunitari, e il recepimento della direttiva 2008/115/CE, e di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. Il provvedimento mira a rispondere a specifici atti dell'Unione europea; infatti, per la libera circolazione dei cittadini comunitari, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per l'incompleto o non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE. Inoltre, la stessa Commissione ha già avviato la fase prodromica all'apertura dell'infrazione per il mancato recepimento della direttiva 2008/115/CE, il cui termine di trasposizione è scaduto il 24 dicembre 2010. Per tale motivo, la sussistenza degli essenziali presupposti di necessità ed urgenza è stata individuata - anche in Commissione affari costituzionali in sede di pronunzia sui presupposti nonché ovviamente dalla relazione illustrativa - nella necessità di evitare le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi dell'Unione europea e nell'urgenza di rispettare le scadenze temporali imposte dalla normativa dell'Unione stessa e dalla disciplina delle procedure d'infrazione. Il decreto-legge, formulato prevalentemente in forma di novella di provvedimenti in vigore, modifica principalmente il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva circolazione dei cittadini comunitari. Viene modificato anche il decreto

le principali modifiche apportate alla disciplina della circolazione dei cittadini dell'Unione europea

che non siano, a loro volta, cittadini dell'Unione europea ai fini del soggiorno fino a tre mesi dell'iscrizione anagrafica, nonché del rilascio della carta di soggiorno di durata superiore a tre mesi. è dato seguito al rilievo mosso dalla Commissione europea, secondo il quale la normativa italiana sovrappone i requisiti per l'ingresso e quelli per il soggiorno, in difformità da quanto previsto da alcuni articoli della citata

Viene poi disposto che ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno oltre i tre mesi deve, in ogni caso, essere valutata la situazione personale complessiva dell'interessato. A tal fine la Camera dei deputati ha stabilito che la verifica si svolga con particolare riguardo alle spese afferenti l'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà, o detenuto in base ad un altro diritto soggettivo. La Commissione europea ha infatti precisato che la direttiva non prevede la quantificazione di un importo minimo prefissato per legge, contenendo solo un generico richiamo ad escludere il ricorso a prestazioni di assistenza sociale. Il decreto legislativo n. 30 del 2007 contiene una norma che fissa importi minimi commisurati all'importo annuo dell'assegno sociale,

Altro punto. La verifica delle condizioni richieste ai fini del mantenimento del diritto di soggiorno potrà essere disposta solo in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime. Si prevede poi che il possesso del documento di attestazione d'iscrizione anagrafica o del documento di soggiorno non costituisca condizione per l'esercizio di un diritto. Questa disposizione è stata modificata dalla Camera dei deputati, che ha introdotto un emendamento diretto ad inserire la parola «necessaria» con riferimento alla condizione. contesto documentale può essere condizione, nei casi previsti dalla legge, per l'esercizio di un diritto, ma generalmente non costituisce condizione per l'esercizio della gran Vengono poi apportate modifiche ai presupposti che possono giustificare l'adozione di provvedimenti limitativi del diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione europea. Si specificano cioè i tradizionali concetti di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza e altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. La minaccia all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza deve essere concreta, effettiva e sufficientemente grave; previgente la minaccia doveva essere solo concreta e attuale. Quindi, si è specificato in modo migliore il concetto di minaccia resta fermo il principio, molto importante, di proporzionalità. Ai fini dell'immediata esecuzione del provvedimento di allontanamento si prevede che l'urgenza sia valutata caso per caso, in relazione all'incompatibilità dell'ulteriore permanenza dell'interessato sul territorio nazionale rispetto al mantenimento della civile e sicura convivenza. L'eventuale ricorso al sistema di assistenza sociale da parte del cittadino dell'Unione europea non potrà essere considerato automaticamente come causa di allontanamento, ma dovrà essere valutato caso sia valutata caso per caso, in relazione all'incompatibilità

si deve poi dimenticare che in caso di inottemperanza al provvedimento di allontanamento, invece della contravvenzione precedentemente prevista, il prefetto, valutato il singolo caso, adotterà un ulteriore provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico immediatamente eseguito dal questore. Viene istituita, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della direttiva n. 38 del 2004, la collaborazione fra Stati membri dell'Unione europea affinché ogni Stato possa, se richiesto, fornire informazioni sui precedenti penali del cittadino o di un suo familiare. La consultazione può avvenire solo per casi specifici ed esigenze concrete. Qui finisce l'esame, molto sommario, della parte che riguarda le modifiche alla direttiva sui cittadini Le principali modifiche apportate al Testo unico sull'immigrazione per dare attuazione alla direttiva sui rimpatri - quindi ciò che riguarda i cittadini extracomunitari - sono le seguenti. Viene introdotto il permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato dal questore. Al fine di incentivare l'esodo volontario dei cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, si prevede che non commetta il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato lo straniero identificato dalla polizia di frontiera in uscita dal territorio nazionale. Viene specificato che l'espulsione di competenza del prefetto sia disposta caso per caso. L'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per mezzo della forza pubblica, che nel testo previgente costituiva la regola generale, viene circoscritta ad una serie di situazioni espressamente individuate. Per tutti gli altri casi si introduce la disciplina della concessione di un termine per la partenza volontaria questo è uno dei punti più nuovi e qualificanti del provvedimento - prevedendo che il questore applichi misure per assicurare l'effettività del provvedimento di allontanamento e stabilendo, in caso di mancato rispetto, una multa da 3.000 a 18.000 euro e l'espulsione. Il meccanismo, più analiticamente, prevede che, salve quelle situazioni espressamente individuate, che continuano a comportare l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione possa chiedere al prefetto la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, che vengono previsti dalla nuova normativa (articolo 14-*ter*). Detto periodo può essere stabilito tra sette e trenta giorni, con possibilità di proroga per ragioni familiari o sociali. Dopo la concessione del termine, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche lecite e proporzionali al termine concesso e dispone altresì una o più delle seguenti misure: consegna del passaporto, da restituire al momento della partenza; obbligo di dimora in un determinato luogo; obbligo di presentazione in giorni ed orari stabiliti presso un ufficio della forza pubblica. Il provvedimento

anni e fino a cinque. Lo straniero potrà d'ora in avanti essere trattenuto nei Centri di identificazione ed espulsione qualora sussistano situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento. Tali situazioni ricomprendono ma non esauriscono - questa è la novità - le cause di trattenimento elencate dalla formulazione previgente, cioè necessità di procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero acquisizione di documenti per il viaggio. Salvo i casi più gravi, sono introdotte misure meno coercitive, alternative al trattenimento nei CIE: consegna del passaporto, obbligo di dimora e obbligo di presentarsi presso un ufficio della forza pubblica. È prevista la convalida del giudice di pace. Il periodo massimo di trattenimento nei CIE è aumentato da sei a diciotto mesi, salvo verifiche della situazione,

Il termine entro il quale lo straniero deve lasciare il territorio nazionale su ordine del questore, qualora non sia stato possibile il trattenimento presso il CIE, è aumentato da cinque a sette giorni. Le sanzioni per l'inottemperanza all'ordine del questore a lasciare il territorio nazionale,

Si prevede poi che la violazione dell'obbligo di espulsione non sia punita qualora sussista un giustificato motivo. Ricorderemo anche in questo caso che vi è stata una sentenza della Corte costituzionale che si era posta questo problema: quando il questore aveva ordinato di allontanarsi dal territorio, il cittadino extracomunitario poteva dimostrare che vi erano una serie di ragioni, la principale quella dei mezzi, che impedivano l'allontanamento e costituivano quindi un giustificato motivo. Da ultimo si prevede che il Ministro dell'interno attui programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza. Si subordina poi l'espulsione o il respingimento delle persone vulnerabili, disabili, anziani, minori e così via alla verifica della loro concreta situazione personale, debitamente accertata. In definitiva, la normativa in esame, in ossequio alle direttive europee, apre a situazioni più morbide senza tralasciare il rispetto della sicurezza.

il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge, cioè l'introduzione, o meglio il tentativo di reintroduzione del limite massimo di trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione per un periodo di 18 mesi. Questa disposizione modifica, come è noto, il comma 5 dell'articolo 14 del Testo unico delle leggi che riguardano e regolano l'immigrazione e la condizione giuridica dello straniero, e lo si giustifica attraverso la necessità di adeguare alla direttiva comunitaria che si occupa del rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi che si trovino in condizione di irregolarità. E questa è la prima ragione per E questa è la prima ragione per la quale viene giustificata la necessità e l'urgenza di fare ricorso, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, al decreto-legge. questa necessità e urgenza non si ravvisa, posto che già la norma in questione prevede un limite massimo di 12 mesi, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE ed il decreto non si limita a recepire la direttiva, ma modifica in modo sostanzialmente innovativo e restrittivo l'ordinamento vigente, peraltro in violazione dell'articolo 4 della direttiva medesima che, quanto alla sua attuazione, garantisce l'operatività e l'efficacia di norme eventuali che già gli ordinamenti nazionali posseggono anche nel caso in cui siano più favorevoli, come nel caso di specie. Da questo punto di vista, emerge già un primo profilo di incostituzionalità della norma che si dice debba essere introdotta con estrema velocità perché così, impone l'Europa. Ma non è così, perché l'Europa dice sostanzialmente una cosa diversa: dice cioè che c'é la necessità di disciplinare,

è sempre relativo a questa disposizione e, segnatamente, alla violazione degli articoli 3 e 13 della Costituzione. Sono, infatti, oggettivamente ed evidentemente violati i princìpi di proporzionalità, di eguaglianza e di adeguatezza nella applicazione applicazione di misure che hanno ad oggetto la restrizione della libertà personale, con riferimento alla sostanziale introduzione di uno stato di detenzione dipendente da una situazione di irregolarità amministrativa. Ricordiamo nel caso specifico il trattenimento per 18 mesi nel Centro di identificazione ed espulsione non segue ad un accertamento della irregolarità o, comunque, della illiceità della permanenza dello straniero nel nostro territorio, ma è solo ed esclusivamente funzionale alla identificazione dello straniero, indipendentemente dal fatto che questo abbia o meno commesso un reato, abbia o meno commesso un illecito amministrativo, si trovi o meno in una condizione di irregolarità. quindi evidente che questa misura è apertamente in contrasto con gli articoli 10 e 13 della Costituzione e lo è ancora di più

privazione temporanea della libertà personale e lo fa anche con riferimento ad ipotesi che riguardano l'immigrazione clandestina, quindi come strumento funzionale al contrasto a tale fenomeno. Ma queste ultime sono ipotesi diverse da quelle che invece vengono disciplinate da questa disposizione. L'articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, infatti, ammette lo stato di detenzione se si tratta dell'arresto o della detenzione regolare di una persona al fine di impedirle di entrare illegalmente nel territorio dello Stato, o contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione.

e che quindi deve essere espulso dal territorio dello Stato: in questo caso, il suo stato di detenzione e la restrizione della libertà personale sono funzionali al suo allontanamento dal territorio nazionale e alla sua espulsione.

(un anno e mezzo) di permanenza all'interno di queste strutture riguarda soggetti che non sono stati colpiti da provvedimenti di espulsione, né sono stati colti nell'atto di entrare illegalmente nel territorio dello Stato. Si tratta di persone il cui stato di regolarità o irregolarità rispetto alle leggi che disciplinano la condizione giuridica dello straniero nel nostro territorio deve essere accertato; pertanto, la misura della detenzione preventiva di 18 mesi è funzionale in via esclusiva alla identificazione del soggetto, e ciò indipendentemente dal fatto che questa persona possa essersi o meno macchiata di una condotta illecita. È evidente che anche da questo punto di vista la norma è incostituzionale, e lo è ancora di più se la paragoniamo alla norma del codice di procedura penale che si occupa del fermo per identificazione, che consiste, com'è noto, nel potere della polizia giudiziaria di trattenere la persona nei cui confronti vengono svolte indagini per il periodo necessario a identificarla. Tuttavia, nonostante si tratti dell'identificazione di un indagato per un reato penale, quindi di un soggetto a cui carico vi possono essere indizi di reato, cioè che abbia avuto delle condotte gravi, l'articolo 349 del codice di procedura penale prevede termini limitatissimi per il suo trattenimento: addirittura, prevede termini così stretti (dodici o ventiquattro ore) da funzionali in via esclusiva alla identificazione del soggetto. Da ultimo, signor Presidente, credo che questa disposizione violi gli articoli 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, perché l'introduzione di un tetto di diciotto mesi per la permanenza in un Centro di identificazione equivale a una condanna ad una pena detentiva senza la commissione di un reato. reato. Guardiamo alla disciplina della custodia cautelare in carcere, e mi rivolgo ai colleghi che sono garantisti a giorni alterni,

in questione soggetti che non si sono macchiati di alcun reato, solo ed esclusivamente al fine della loro identificazione. Faccio qualche esempio, così ci comprendiamo e comprendete. Tutti i reati puniti con la reclusione non inferiore a vent'anni (associazione mafiosa, reati aggravati da metodo mafioso, delitti di terrorismo e eversione, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, delitti in materia di armi, spaccio di sostanze stupefacenti, reati di pedopornografia e violenza sessuale) prevedono un limite massimo della custodia cautelare in carcere di Voi per i mafiosi prevedete un massimo di dodici mesi di custodia cautelare; per lo straniero, che non si sa se regolare o irregolare perché deve essere accertato, prevedete diciotto mesi di detenzione in un Centro di identificazione ed espulsione. con cui pensate di affrontare un tema complesso e delicato come quello del contrasto all'immigrazione clandestina, c'è obiettivamente da mettersi le mani nei capelli, c'è obiettivamente da indignarsi. Peraltro, in questi anni non avete costruito nuovi Centri di identificazione ed espulsione, sono sempre quelli, anzi, forse qualcuno è stato pure chiuso,

di assoluto disagio; tutto questo determinerà ciò che in parte si sta già determinando in parecchi Centri di identificazione, cioè i disordini e l'abbandono, cui si risponde, come è stato ad esempio per i fatti di ieri e oggi, istigando la polizia - anche dal giornale della Lega - a sparare su persone che chiedono di sapere qual è la loro condizione rispetto alla legge che disciplina la condizione giuridica dello straniero. Questa è una norma da incivili, oltre che incostituzionale, di cui vi dovete vergognare.

Signor Presidente, credo che si debba innanzitutto premettere che, a dispetto della straordinaria necessità ed urgenza richieste dall'articolo 77 della Costituzione, esiste, in particolare in questa legislatura, un tasso di decretazione d'urgenza che rasenta l'abuso. Quali garanzie, allora, per la legalità costituzionale e per i cittadini? Ma, soprattutto, a quale funzione strutturale nell'azione di Governo risponde oggi il decreto-legge? Quanto all'emergenza, l'immigrazione clandestina non è un fenomeno nuovo, né imprevisto. L'emergenza risiede invece nel modo in cui le problematiche inerenti l'immigrazione clandestina sono state gestite dal Governo, ma questo certo non rientra nei postulati dell'articolo 77 della Costituzione. La gestione emergenziale tradisce dunque, in primo luogo, una reazione irrazionale da parte del Governo e testimonia la fragilità di di un Esecutivo che tenta di governare malgrado il Parlamento. Sfortunatamente, «governare malgrado il Parlamento» non è esattamente l'idea che ci facciamo di una democrazia parlamentare. C'è dunque una vera necessita?

ed urgenza che sono richiesti dall'articolo 77 della Costituzione? Senza delegazione delle Camere il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge. Il rischio maggiore di un Parlamento che non riesce a legiferare è che pone le condizioni oggettive di legittimazione del suo aggiramento o commissariamento, secondo un'interpretazione che la Costituzione concede

valore di legge. Il rischio maggiore di un Parlamento che non riesce a legiferare è che pone le condizioni oggettive di legittimazione del suo aggiramento o commissariamento, secondo un'interpretazione

Questo processo non è indolore e miete le sue vittime - in questo caso minoranze d'immigrati, ancorché irregolari - ancora una volta sottratte all'imperio giusto del diritto, e gettate nell'abisso dell'eccezione.

un massimo di 18 mesi. La previsione di un prolungato trattenimento non è infatti richiesta obbligatoriamente dalla direttiva rimpatri, ma è prevista come facoltà concessa agli Stati membri. Ci sembra quindi che la previsione di questo ulteriore termine sia di natura meramente formale e serva soltanto a rassicurare l'opinione pubblica sulla volontà del Governo di assicurare una gestione rigorosa degli ingressi nel territorio nazionale. Va ricordato che con il pacchetto sicurezza l'Italia aveva già aumentato questo periodo da due a sei mesi dalle statistiche dello stesso Viminale sappiamo che in pochissimi casi chi non può essere espulso in due mesi potrà esserlo in sei. Ora, portarlo a 18 mesi è solo una punizione una punizione che non ha nulla a che vedere con una vera politica di rimpatri, perché non cambia l'effettività dell'allontanamento della persona dal territorio. È quindi solo un atto punitivo, considerate le condizioni in cui versano questi Centri. L'estensione dalla durata massima è ancora più preoccupante quando avvenga senza che siano previsti un rafforzamento delle garanzie e dei diritti dei soggetti trattenuti e un adeguamento delle condizioni dei CIE e dei relativi servizi. Dato che il CIE esiste ai fini dell'espulsione, se questa non può realizzarsi, la reclusione perde la sua ragione d'essere: esattamente quanto prevede la direttiva n. 115 del 2008, quando introduce una gradazione di provvedimenti da prendere Mi sento, infine, di sottolineare un aspetto di carattere generale: si sta enucleando un diritto della cittadinanza europea applicato ai cittadini dell'Unione e ai cittadini extracomunitari. Le questioni sono complesse e - ci rendiamo conto - anche difficili da risolvere tecnicamente. conto - anche difficili da risolvere tecnicamente. Mi pare che il Governo si sia mosso entro una cornice molto stretta: pur rispettando formalmente il dato europeo delle direttive, ha tuttavia accolto un'interpretazione eccessivamente estesa delle facoltà concesse agli Stati membri. Credo, piuttosto, che su tali questioni vada aperto un raccordo permanente con la Commissione europea: che intervenire con decreti come quello oggi al nostro esame, ciò consentirebbe di prevenire l'insorgere di procedure di infrazione o - peggio - di sentenze come quella sulla clandestinità, che sicuramente non rafforzano l'immagine italiana a livello europeo.

Penso poi alla disuguaglianza, nonostante gli articoli 3 e 13 della Costituzione parlino di proporzionalità, uguaglianza e adeguatezza nell'applicazione. Si pensi anche al fermo previsto dal codice di procedura penale per colui che è sospettato di aver commesso un reato e che non possa essere identificato:

alla detenzione di un anno e mezzo, c'è da rabbrividire, soprattutto perché la Costituzione è stata completamento dimenticata. CIE. Voi vivete lontani dalla realtà. Questo è semplicemente uno scambio di provvedimenti: io do un processo lungo a te e

La verità non è quella secondo cui occorre un anno e mezzo per identificare una persona. Chiunque sa che se la persona non viene identificata in 15 giorni, in un mese, in tre mesi, in tre mesi, non è possibile poi identificarla in un anno e mezzo. Allora, al termine dell'anno e mezzo verrà messo un foglio in mano all'immigrato e gli sarà detto che ha dieci giorni per lasciare il nostro Paese. A me sembra che questa non sia civiltà: a me sembra che siamo lontani dall'Europa. Pensiamo di farci apprezzare dall'Europa e poniamo in essere un provvedimento assolutamente illegittimo, assolutamente contrario alla nostra Costituzione. Com'è possibile non rendersi conto di quello che sta avvenendo nel nostro Paese? Io condanno la violenza di quegli stranieri che ieri hanno occupato l'autostrada, ma come non si può comprendere la rabbia di questa gente, la rabbia di persone che aspettano di essere ammesse all'asilo, e questa attivazione da parte dello Stato non Allora si occupano le autostrade, si occupano le ferrovie. Siete lontani dalla realtà. Bisogna tener presente qual è l'obiettivo reale. L'obiettivo reale di questo provvedimento non è di identificare in un anno e mezzo i cittadini stranieri, ma è quello di scoraggiare l'ingresso nel nostro Paese. Questa non è politica: questa non è la politica che il sottoscritto e il nostro Gruppo intendono seguire.

pregiudiziale ed esporre una considerazione che riguarda il Capo II, cioè la direttiva rimpatri per la parte che attiene ai cittadini extracomunitari,

dobbiamo tutti chiarirci, perché c'è un equivoco per chi non ha analizzato attentamente il provvedimento. La direttiva contiene una serie di misure, anche piuttosto analitiche, che hanno imposto la revisione perché saremmo già in procedura di infrazione. Contiene anche il riferimento all'anno e mezzo, ma non è su questo che l'Italia è in violazione: è in violazione sulle altre procedure.

non è una norma in contrasto con la direttiva. Quindi, prego tutti di non ripetere che bisogna stabilire l'anno e mezzo perché ce lo chiede la direttiva. Non è così, è una menzogna, e dobbiamo smetterla di trasmettere all'esterno questa menzogna. Il Parlamento italiano ha deciso che il proprio termine per il trattenimento nei CIE è di sei mesi, e in questo non è per nulla in contrasto con la direttiva. Quindi, questa misura non andava toccata attraverso un provvedimento di necessità e urgenza, la cui necessità e urgenza deriva solo dall'esigenza di applicare la direttiva e non essere difformi. Questa parte, se vogliamo procedere

motivata solo da circostanze estranee alla condotta individuale - quali l'indisponibilità dei documenti di viaggio o l'impossibilità di identificare lo straniero, non già la sua resistenza all'identificazione rischia di contrastare non solo con il principio di ragionevolezza, ma anche con la stessa direttiva, pur invocata dal Governo a sostegno della normativa. Dal punto di Dal punto di vista della direttiva comunitaria, il decreto‑legge contrasta con la recente interpretazione della direttiva stessa data dalla Corte di giustizia dell'UE nella sentenza del 28 aprile 2001 (caso El Dridi, che è stato è stato riportato ampiamente nelle cronache), nella quale la Corte ricorda che la successione delle fasi della procedura di rimpatrio dello straniero in condizione di soggiorno irregolare stabilita dalla direttiva corrisponde ad una gradazione delle misure da prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio. In altre parole, l'espulsione è l'ultima delle misure attivabili. Essa, infatti, appare strettamente regolamentata nella direttiva «allo «allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini interessati dei Paesi terzi (...): il principio di proporzionalità esige che il trattenimento di una persona sottoposta a procedura di espulsione o di estradizione o di estradizione non si protragga oltre un termine ragionevole, cioè non superi cioè il tempo necessario per raggiungere lo scopo perseguito. Secondo tale principio, il trattenimento ai fini dell'allontanamento deve essere quanto più breve possibile». Il Parlamento

cui, avendo dovuto recepire per forza la direttiva, perché altrimenti tutti i tribunali italiani non avrebbero più ratificato i provvedimenti di pubblica sicurezza, lei approfitti di questo testo per ritornare sull'anno e mezzo che questa Camera le ha bocciato.

Il profilo chiaramente più evidente è quello del difetto previsto all'articolo 77 della Costituzione, ossia il carattere di urgenza dell'attuale decreto. Si introduce con il decreto una disciplina estremamente particolare, che basterebbe leggere nella sua articolazione per rendersi conto della sua assurdità. La permanenza nei Centri di accoglienza e di espulsione può essere prorogata fino a 30 giorni; trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di 60 giorni. Quando persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di 60 giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per periodi non superiori ai 60 giorni, fino a un termine massimo di ulteriori 12 mesi. questa gradualità di allungamento della permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione è contraria a un criterio di ragionevolezza ed è in violazione anche con il principio della previsione di durata di misure amministrative, quale essa è. Anche se di natura amministrativa, è sempre privazione della libertà personale, non può prevedersi la durata di una misura amministrativa di privazione della libertà personale non ancorata a un comportamento, ma ad una ad una non collaborazione da parte degli Stati che dovrebbero facilitare l'identificazione del soggetto. Ossia, la permanenza nel Centro di identificazione da 30 giorni può arrivare a 18 mesi non per il comportamento del soggetto, ma perché uno Stato non collabora a fornire i dati per procedere all'identificazione. Mi sembra, francamente, che una previsione di questo genere vada al di là di ogni criterio di ragionevolezza, perché incide sullo *status* di libertà di una persona, non per fatto attribuibile alla persona stessa, ma per fatto che dipende dall'inerzia dall'inerzia amministrativa di nostri uffici o degli uffici richiesti. Non si può affermare che si resta perché si è tardato nell'inoltrare la pratica amministrativa o perché chi doveva rispondere ancora non ha risposto. In discussione non è una pratica amministrativa. In discussione è la libertà della persona. È questo il contrasto profondo con i nostri principi costituzionali, come, nel nostro sistema processuale, le misure cautelari siano restrittive della libertà personale, siano progressive ma con un limite massimo, arrivando ad un anno per i reati più gravi, prevedendosi in alcuni casi delle specifiche proroghe ma, comunque, sempre limitate. Qui, invece, stiamo andando a delle proroghe esorbitanti, e non per un fatto attribuibile ad un soggetto, ma per un fatto esterno alla volontà del soggetto. La libertà personale è un bene assoluto, e noi non possiamo farlo diventare materia di gestione amministrativa. L'assolutezza del principio della libertà personale non è pratica amministrativa, ma appartiene alla categoria dei diritti assoluti. E in questo c'è il profondo contrasto con i principi della nostra Costituzione, della quale noi andiamo orgogliosi:

che il termine massimo di detenzione in questi Centri può essere di 12 mesi, salvo deroga più favorevole da parte degli Stati.

Signor Presidente, la conversione di questo decreto-legge sul recepimento della direttiva europea sui rimpatri merita alcune considerazioni generali, relative all'incapacità di questo Governo di guidare ancora il Paese. Se infatti ci soffermiamo, come esempio paradigmatico, sul metodo utilizzato per portare avanti il recepimento di tale direttiva, vediamo come esso sia caratterizzato da palesi confusioni e contraddizioni. Infatti, nel 2008, si avviò il procedimento di recepimento della direttiva, poi insabbiato dal PdL,

avviene solo nel caso in cui la normativa nazionale sia in qualche modo più favorevole dell'ordinamento europeo: e non è così, per quanto riguarda il nostro Paese. Ebbene, in questo stato confusionale di ritardi e di incertezze, avete prodotto nell'azione di Governo un grave ritardo rispetto all'Unione europea, da dover adottare un decreto-legge per giustificare l'urgenza di un Governo confuso, che complica la vita a se stesso e al Paese. Veniamo poi al merito del provvedimento, che dimostra il vostro fallimento e la vostra inadeguatezza almeno sotto quattro profili: nel rapporto con l'Europa, per quanto riguarda il quadro delle norme comunitarie; sul piano economico, per quanto riguarda un attento utilizzo delle risorse, ancora deficitarie; sulla sicurezza; sull'immigrazione. Infatti, rispetto al rapporto con l'Europa è ben chiaro che sul tema dell'immigrazione non avete fatto brillare l'Italia per comportamenti virtuosi e avete dimostrato le contraddizioni politiche di una maggioranza che, apparentemente, non ha assolutamente avuto la capacità di recepire adeguatamente la normativa e, al tempo stesso, è in contraddizione per quanto riguarda il partito di maggioranza con l'atteggiamento che il PPE ha avuto nel Parlamento europeo. In un contesto quindi di rapporti già delicati con l'Unione europea, dovuti alla gravità dei fenomeni sull'immigrazione l'Italia per bocca dei suoi Ministri più volte si è distanziata dal percorso condiviso dagli altri *partner*. Se a ciò aggiungiamo le difficoltà giudiziarie e scandalistiche che hanno attraversato la vita di questo Governo, ci rendiamo conto di quanto sia fragile e poco autorevole la nostra iniziativa in campo europeo. Inoltre, il provvedimento non è per niente rispettoso del quadro comunitario relativamente soprattutto ai trattenimenti nei e anche in relazione alle disposizioni circa a necessità - ci ricorda la direttiva europea - di adottare misure invece via via più proporzionate e più intense, e cioè di preferire lo strumento del rimpatrio volontario come misura prioritaria. Al contrario, abbiamo la sensazione che in questo provvedimento, per il combinato disposto delle norme stesse e di quelle da noi adottate già in precedenza, da questo Governo proposte sulla sicurezza, ci troviamo di fronte ad una dissuasione dei rimpatri volontari. Pensiamo, per esempio, ai ritardi relativamente alla documentazione che possono essere non di responsabilità dell'immigrato o all'impossibilità di dimostrare l'alloggio per le disposizioni che ricordiamo sulla sicurezza che potrebbero colpire il locatario. In sostanza, il combinato disposto di queste norme dissuade e voi ottusamente perseguite, in contrasto con la stessa normativa e rischiando ulteriori sanzioni, il ricorso ai CIE. Se esaminiamo anche le sentenze della Corte di giustizia, ci dobbiamo preoccupare per la futura evoluzione, in quanto è stato affermato che i giudici degli Stati membri sono tenuti a disapplicare norme interne che siano in contrasto con la direttiva e ad applicare direttamente quelle della direttiva stessa. Quindi, non siamo sereni circa i futuri esiti di questo stesso recepimento. Per chiudere il contenzioso con l'Unione europea, abbiamo perciò proposto numerosi emendamenti anche alla Camera, che avete respinto, attivando ancora una volta un atteggiamento di chiusura, e non credo a favore del nostro Paese. Con il decreto-legge in esame violate gli impegni che l'Italia aveva assunto a Bruxelles, perché in fondo la permanenza nei CIE - dobbiamo dirlo - diventa una forma di reclusione nascosta e di privazione della libertà personale che dovrebbe rappresentare una eccezionalità.

Veniamo alle questioni economiche. L'impatto di questo provvedimento, ossia la permanenza nei CIE, potrebbe far lievitare fortemente i costi. È stato stimato che il costo di tale operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 30.000 euro per 18 mesi per ogni soggetto trattenuto; per non parlare dei costi aggiuntivi in termini di controllo del territorio e dell'ordine pubblico ogni qual volta, proprio per l'esasperazione di questa misura, per il sovraffollamento di tali Centri, si possono creare nei luoghi circostanti

una situazione che voi stessi avete contribuito con questo provvedimento ad esasperare, ad aggravare e a rendere meno governabile. Veniamo infine alle questioni relative all'immigrazione e alla sicurezza, a partire dalla legge Bossi-Fini che da tempo doveva essere rivista per le sue notevoli incongruenze e fallimenti, incapace di gestire una politica migratoria ordinaria, figuriamoci una politica migratoria aggravata dai contesti e dai conflitti internazionali e dalle condizioni che l'altra sponda del Mediterraneo sta vivendo. Se a questo provvedimento si aggiungono quelli già adottati sulla sicurezza e la vostra ossessione di scaricare sull'immigrazione tutte le paure, le insicurezze e gli eventi criminali, la cifra della capacità di governare i problemi complessi si abbassa di molto perché essa richiederebbe invece ascolto, confronto, ricerca di soluzioni possibili in contesti difficili, arte del governo a cui - pare - non siate molto allenati,

la tragedia di Lampedusa, gli scontri con gli extracomunitari del Centro di accoglienza di Bari, la ripresa degli sbarchi e le continue morti non ci fanno stare tranquilli.

L'intesa con la Tunisia funziona grazie all'accordo che il ministro Maroni ha sottoscritto: e i flussi dalla Tunisia sono diminuiti rispetto a qualche mese fa. Con la Libia non riusciamo a stipulare accordi a causa della guerra, ma non possiamo più tollerare questi massacri.

importante. In questi mesi abbiamo affrontato il fenomeno da soli: siamo rimasti da soli. Non possiamo più tollerare una situazione del genere. Cari colleghi, mi dispiace dirlo, ma se non troviamo la giusta soluzione, diventiamo complici dei trafficanti di carne umana, che in questo momento stanno studiando

le forze dell'ordine di Lampedusa e i vigili del fuoco, che ieri hanno fatto un lavoro straordinario (sono riusciti

cari colleghi, non può affrontare un massacro del genere. È un piccolo fazzoletto di isola, è una terra che ha bisogno di stare tranquilla. Abbiamo bisogno tutti di vedere il nostro Paese in modo sereno e diverso, e non è giusto che critichiamo chi vuole fermare questi massacri. In qualche modo li dobbiamo fermare. Caro Ministro, vorrei farle i complimenti per il lavoro svolto in questi anni, ma abbiamo bisogno di risposte serie, perché né Lampedusa né il nostro Paese possono più tollerare una situazione del genere.

In effetti va detto che, a parte il ritardo di quasi otto mesi relativamente al recepimento della direttiva europea sui rimpatri, il Governo ha modificato le proprie politiche. Si è infatti passati dall'eclatante respingimento, contro tutti i diritti umani codificati da cinquant'anni a questa parte, alla creazione di una nuova linea di bilancio per il nostro Stato, cioè il sostegno vitale a chi scappa da zone colpite da carestie, guerre e incertezze. Si è creato un ottimo sistema economico, quello dei Centri di prima accoglienza, dei Centri di accoglienza ai richiedenti asilo, dei Centri di identificazione ed espulsione. Secondo il Ministero dell'interno, saremmo capaci di dare ospitalità - con tutte le virgolette del caso - a circa 7.650 persone,

Per quattro anni, incluso il decreto che ha ancora una volta commissariato questo regime antidemocratico che passa alla storia come Repubblica italiana, erano già stati, in deroga a tutte le normative nazionali e internazionali, stanziati 10 milioni per le prime tendopoli di accoglienza dei flussi dell'emergenza migratoria dal Nord Africa. Con quanto andiamo a votare oggi, verranno stanziati ulteriori 16.824.813 euro

circa 5.000-6.000 persone per i prossimi quattro anni, contro tutti i trattati internazionali riconosciuti dall'Italia, ma in virtù dei poteri dati al commissario straordinario, uno degli 8.000 che esistono oggi in Italia per la gestione e - ahimè! - non il governo del fenomeno, essendo egli capace di poter prendere decisioni in deroga a qualsiasi normativa.

l'assistenza a queste persone. mandato all'interno di questi Centri (magari se si è della maggioranza o del Governo è meglio entrarci sotto mentite spoglie perché l'accoglienza potrebbe non essere delle più favorevoli). iniziare a girare luogo per luogo per controllare la qualità delle strutture, e soprattutto per trovare il modo migliore per comunicare a chi oggi vi è recluso che dai 6 mesi massimi di trattenimento si passerà ad un anno e mezzo. sicuramente ciò che è avvenuto ieri a Bari ed a Crotone sarà la norma, da stanotte, quando cioè questo decreto diventerà legge, perché sicuramente non verrà accolto nel migliore dei modi da chi scappa da violenze, persecuzioni, carestia e morte, proprio come scappavano magari gli italiani 150 anni fa. negli ultimi giorni le discussioni sui provvedimenti all'attenzione di quest'Assemblea sono state caratterizzate da due costanti: la prima è la richiesta a quest'Assemblea di convertire un decreto d'urgenza, e di convertirlo in tempi strettissimi, senza quindi la possibilità di entrare, come si dovrebbe, nel merito del provvedimento; un provvedimento per il quale, tra l'altro, il ricorso alla decretazione d'urgenza da parte del Governo rappresenta ancora una volta un'anomalia da superare. Il secondo dato, che in parte forse spiega anche il primo, è che ancora una volta, dietro questo provvedimento, si annida la volontà, o la necessità, di una forza politica della maggioranza di ricavarne in questo momento uno strumento di demagogia e di propaganda. E questo mi dispiace. Ciò, a dispetto, e purtroppo a discapito, di un tema delicatissimo, come quello dell'immigrazione, per il quale il nostro Paese è già incappato in una procedura di infrazione europea, come hanno detto altri colleghi. Voglio ricordare che proprio la settimana scorsa ci trovavamo in quest'Aula chiamati anche in quel caso a convertire un decreto-legge d'urgenza, anche in quel caso su una materia estremamente delicata, quale l'autorizzazione e il finanziamento delle missioni italiane all'estero, sulla quale il reiterato ricorso alla decretazione d'urgenza era stato più volte, anche in passato, giudicato inappropriato, sia dalle forze dell'opposizione sia da esponenti della maggioranza. E anche in quel caso qualcuno ne ha approfittato per fare demagogia a spese dell'immagine dell'Italia all'estero: gli stessi che allora hanno parlato di *exit strategy*, in modo assolutamente inappropriato e completamente fuori luogo rispetto alle priorità e alla linea di politica estera del Paese, oggi colgono l'occasione per mostrare ai propri elettori che fanno passare la linea dura nei confronti dell'immigrazione. Per questi motivi di ordine generale, sui quali non mi soffermerò oltre, ancora una volta le Commissioni non sono state poste nella condizione di esaminare il provvedimento per tempo e, soprattutto, con sufficiente tempo a disposizione. E voglio solo ricordare i punti di maggiore criticità, sui quali sarebbe stato più che mai opportuno un approfondimento delle nuove norme in sede parlamentare. Solo un esame più attento dell'intera materia avrebbe assicurato il superamento *in toto* delle pregiudiziali che hanno fatto incorrere l'Italia nel procedimento di infrazione in sede europea e che in queste condizioni invece io non sarei certa di poter definire completamente superate. all'allungamento da 6 a 18 mesi del trattenimento presso i Centri di identificazione ed espulsione, voglio ricordare che la direttiva europea prevedeva questo termine come un fatto da applicare in condizioni assolutamente straordinarie, e non per trasformare i CIE in luoghi dove in luoghi dove le persone vengono di fatto private della libertà per 18 mesi. Le persone non sono semplicemente dei numeri: un anno e mezzo di vita è moltissimo tempo, lo è anche per una persona giovane, non lo dimentichiamo. In tema di rimpatri, nonostante le modifiche apportate da questo decreto-legge alla normativa preesistente, l'espulsione attraverso l'accompagnamento alla frontiera rimane la regola e il rimpatrio volontario rimane l'eccezione. Mentre lo spirito della direttiva comunitaria era esattamente l'opposto. Ciò che secondo me deve essere superato è il criterio a cui si ispira questo, come altri precedenti provvedimenti di questo Governo in tema di immigrazione, e cioè che esiste un *trade off* tra i diritti degli immigrati e le esigenze di sicurezza del nostro Paese e dei nostri concittadini. E invece si propone solo una visione limitata e contingente. Credo che, in una prospettiva di largo respiro, una politica che voglia veramente guardare al futuro debba superare questa visione e cominciare a cercare le complementarità e le sinergie invece che soltanto i *trade off* (per chi lo capisce). Per chiudere, questo è un tema che non può essere trattato con piccoli aggiustamenti e poi rimesso nel cassetto. Il fenomeno dell'immigrazione è in continua espansione e in continua evoluzione e come tale va trattato, con norme che esprimano la lungimiranza della classe politica (non questa) di un Paese, che tra l'altro si muove in un contesto di politica europea dell'immigrazione. Non è cosa da trattare con una leggina, i cui soli risultati sono il tamponamento di alcune falle che si erano aperte sul fronte europeo, e in realtà Soprattutto non dovrebbe essere materia da utilizzare per fare cassa, con un banale risultato di propaganda demagogica.

è stata approvata nel 2008: sono quindi tre anni che il Governo, questo Governo, che ha la delega totale per il recepimento del diritto comunitario, tenta di aggirare ancora oggi l'obbligo del recepimento conforme. Tre anni scanditi da aperture di procedure di infrazione, richiami e richieste di chiarimento da parte della Commissione europea, fino alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che invita i giudici italiani a non applicare le norme nazionali in quanto non conformi al diritto europeo, diritto che ormai, per alcune materie che si riferiscono alla Carta dei diritti fondamentali, è direttamente e immediatamente applicabile. Vedete, la strana schizofrenia che ha improntato l'azione di questo Governo ha portato a discutere nel corso di questi tre anni di restrizione alla libera circolazione dei cittadini comunitari, di preclusione del diritto di matrimonio per gli stranieri irregolari, di respingimento alla frontiera o in alto mare, di reato di immigrazione clandestina, di restrizione al ricongiungimento familiare, di rimpatrio di minori che esercitano la prostituzione e naturalmente di controllo sociale, presidio del territorio da parte delle ronde, di estensione della obbligatorietà della custodia cautelare e di registro dei senza dimora. Nonostante l'imponente pacchetto di misure a tutto campo che l'Unione Europea ha varato in materia di immigrazione, mai abbiamo discusso in quest'Aula un piano organico di regole, diritti diritti e doveri cui conformarsi, tanto da parte degli immigrati quanto da parte dello Stato italiano. Aggiungo che, trattandosi di materia estremamente complessa, che ha intrecci e ricadute con molte altre politiche europee e nazionali, ci sarebbe bisogno di uno sforzo di coerenza e lungimiranza. Vedete, tagliare i fondi della cooperazione allo sviluppo ha ovviamente una ricaduta sui flussi migratori; tagliare i fondi al volontariato nelle missioni internazionali ha una sua ricaduta; tagliare il *welfare* e gli investimenti per il lavoro e la crescita nazionale ha anch'esso una sua ricaduta. E così il problema dell'immigrazione si riduce per questo Governo e questa maggioranza ad un problema esclusivamente di ordine pubblico e sicurezza, alimentando così la deriva negativa e non trovando soluzione nemmeno ai problemi del cosiddetto ordine pubblico. allora ricordare che i dati dei rimpatri effettuati sono fermi al 2009, caro ministro Maroni: non ci fornite mai i dati delle espulsioni e dei rimpatri: perché? Anzi, avete un modo molto singolare di agire: quando dovete accogliere gli immigrati, accompagnate l'accoglienza con l'annuncio di un certo numero di persone respinte, ma i dati sulle persone che trattenete nei CIE e che sono poi davvero respinte sono fermi al 2009, perché sono dati imbarazzanti voi: confermano che non è vero che più lungo è il trattenimento nei CIE, maggiore il numero delle persone rimpatriate. Dunque, ciò che conta non è la durata del trattenimento, che la direttiva stessa prevede in diciotto mesi come ultima*ratio*, e sicuramente non per trattenimenti trattenimenti di massa, ma le altre politiche, a partire da quelle sulla stabilità del Mediterraneo e dalla collaborazione con i Paesi da cui provengono le persone. Se non c'è questa cooperazione e visione globale del fenomeno, potete trattenere le persone anche diciotto mesi, ma dopo non vi resterà altro da fare che dichiarare il fallimento, perché la politica sull'immigrazione che avete scelto di perseguire è costosa, inefficace e disumana, come d'altronde è costosa e farraginosa la procedura di recepimento del diritto comunitario che contraddistingue il nostro Paese. sembra uno scherzo del destino, ma mentre nelle Commissioni 1a e 14a è all'esame un testo per rafforzare la delega al Governo in materia di recepimento del diritto comunitario, di fatto oggi, con tutti i suoi difetti certamente, ci troviamo ad effettuare un recepimento trasparente e coinvolgente: non una delega totale e al buio al Governo, ma un provvedimento su cui il Parlamento si misura e si esprime. È una procedura conforme al nostro sistema parlamentare, che, da una parte, prevede prevede il recepimento e, dall'altra, contestualmente, le modifiche all'ordinamento nazionale; una procedura che rispetta le prerogative dell'Esecutivo e del Parlamento e, allo stesso tempo, assicura semplificazione, trasparenza ed efficienza, almeno le dovrebbe assicurare se vi fosse una residua volontà politica da parte di questa maggioranza di cominciare a lavorare per l'Italia e non più esclusivamente per conservare o conquistare un consenso in chiave populista e demagogica (peraltro anche questo è un risultato mancato, mancato, perché il vostro populismo evoca angosce e fantasmi che poi non è in grado di governare). Appare sempre più evidente la necessità che si sviluppi in ambito nazionale una coscienza più forte della centralità dell'Europa e delle politiche comunitarie. In questo senso, voglio sottolineare che il pacchetto di direttive che regola diritti e doveri degli immigrati negli Stati membri ha visto la partecipazione viva ed attiva del Governo italiano. Mi riferisco, nello specifico, anche alle dichiarazioni del ministro Frattini, che ha sottolineato più volte come per combattere l'immigrazione illegale bisogna dotarsi - e cito - «di un approccio che abbraccia diversi aspetti dell'articolato fenomeno migratorio: politiche di contrasto all'immigrazione illegale; politiche di cooperazione con i Paesi terzi; politiche che permettono agli immigrati di accedere al mercato del lavoro europeo, dove tante professionalità sono già perdute o in via di estinzione;

nella recente risoluzione Pisanu votata qualche mese fa in quest'Aula, noi ci stiamo. E allora, se è questo l'impianto che voi volete, siamo pronti a votarlo, ma ci vuole anche una dimostrazione da parte della maggioranza e, soprattutto, da parte del Governo: accogliete i nostri emendamenti,

Signor Presidente, gentile ministro Maroni, colleghi senatori, oggi diamo un chiaro segnale di continuità e di coerenza, messo in atto dalla Lega Nord e dal Governo, capace di recepire, interpretare e far proprie le finalità della direttiva volta ad istituire «un'efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della loro dignità». Vorrei subito ricordare, soprattutto ai colleghi dell'opposizione, che questo decreto si è reso necessario per evitare le procedure di infrazione comunitaria per l'incompleto e non corretto recepimento delle direttive europee sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e sul rimpatrio dei clandestini. La Lega Nord, e in particolare il ministro Maroni, ha quindi seguito il principio del buonsenso, dando applicazione a normative che già esistono. Non si tratta di razzismo, xenofobia o di caccia all'uomo nero, come spesso qualcuno - soprattutto tra i colleghi dell'opposizione - ci accusa. Chi viene nel nostro Paese con un serio progetto di vita è una risorsa, ma oggi non possiamo più

immigrazione dopo le rivolte in Tunisia che, com'è stato detto, sono state risolte grazie agli accordi, anche se adesso la guerra in Libia sta determinando una situazione assolutamente insostenibile. Al riguardo, ritengo che sia opportuno, come abbiamo già fatto ieri, esprimere la nostra solidarietà alle forze dell'ordine che sono state coinvolte negli scontri con gli immigrati. Ma torniamo al merito del provvedimento, per fare un esempio dell'ampia condivisione di questo documento, vorrei citare il parere dell'Alta Commissione delle Unite per i rifugiati, che si è espressa in modo positivo in merito all'introduzione nell'ordinamento italiano, nel contesto, quindi, del recepimento, della direttiva rimpatri, del cosiddetto rimpatrio volontario assistito, cui possono accedere anche persone e situazioni irregolari e persone colpite da provvedimento di respingimento o di espulsione. La stessa Commissione, poi, ha accolto con favore il fatto che i richiedenti asilo ai quali non è stata riconosciuta nessuna forma di protezione, abbiano l'opportunità di rimpatriare con modalità che siano rispettose della dignità e della sicurezza della persona, beneficiando, appunto, di programmi di rimpatrio volontario e assistito. Può essere interpretato come meglio si crede, amici dell'opposizione, ma questo decreto-legge pone davvero l'accento sul trattamento delle categorie vulnerabili, che risulta quindi un ulteriore elemento positivo. Potrei commentare questo decreto-legge partendo dal punto fermo, tanto caro al movimento che rappresento in quest'Aula oggi, dello straniero clandestino che deve essere rimpatriato. Lo dice la parola stessa: clandestino, ovvero una persona straniera che si reca in un altro territorio, in violazione delle leggi di immigrazione del Paese di destinazione. Dovremmo quindi accogliere chiunque, dovremmo garantire loro assistenza, lavoro, sostentamento e - magari - anche una casa con tutte le comodità della nostra epoca? Non sarò io a dare la risposta a queste domande, ma lascio rispondere al tempo e ai cittadini, alla gente che

hanno modo e titolo di restare nel nostro Paese, si analizzeranno tutte le varie possibilità: dalla partenza volontaria alle misure coercitive, tenendo presente anche eventuali cause ostative alla partenza volontaria e così via. Su richiesta, quindi, dell'interessato, dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera, resta la possibilità di chiedere al prefetto, ai fini dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario e assistito. Il prefetto, quindi, termine che può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale (quali la durata del soggiorno sul territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola o di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario e assistito). Con questo decreto è stato introdotto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui possono beneficiare anche i minori stranieri non accompagnati, affidati, ovvero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi a un progetto di integrazione sociale e civile. Mi sembra chiaro, quindi, che questo decreto‑legge sia finalizzato, nel suo complesso, a dare attuazione al diritto europeo in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. Come è già stato specificato ed emerso nella discussione alla Camera, il provvedimento che stiamo per adottare nasce in relazione alla straordinarietà e all'urgenza dell'intervento normativo, che si configura come atto obbligatorio per gli impegni assunti dall'Italia in sede europea. Per quanto riguarda l'estensione a 18 mesi del periodo di trattenimento nei CIE, ritengo esso sia un provvedimento necessario al fine di riconoscere i clandestini per poi rispedirli a casa, visto che nessuno di noi vuole mantenerli a spese dello Stato, con vitto e alloggio. Fatichiamo a dare un lavoro alla nostra gente, ad aiutare la nostra gente, provata dalla crisi economica che ancora rallenta la nostra economia. Per questo non dobbiamo illudere nessuno. Il nostro non è il Paese dei balocchi: non si trovano pane, casa, lavoro semplicemente attraccando con un gommone. Purtroppo, già chi è nato e cresciuto nel nostro territorio talvolta non riesce ad arrivare a fine mese, e noi non possiamo più permetterci di star qui a pensare ad aiutare gli ultimi arrivati, dimenticandoci di chi aveva un lavoro, ha pagato i contributi e deve ora persino sobbarcarsi il costo di soggiorno degli ultimi arrivati. In questo decreto anche l'ordine pubblico riveste la sua importanza: per la prima volta, infatti, è prevista l'espulsione dei cittadini comunitari - ribadisco: comunitari - per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Questi, se permangono sul territorio nazionale in violazione delle prescrizioni della direttiva sulla libera circolazione, dovranno lasciare immediatamente il nostro territorio. Mi sembra poi doveroso ricordare anche che con questo decreto-legge l'espulsione sarà immediata in caso di pericolosità dello straniero, mancata richiesta di concessione del termine per la partenza volontaria, inosservanza - senza giustificato motivo - del termine già concesso allo straniero per la partenza volontaria o inosservanza anche di una sola delle misure coercitive applicate nei confronti del cittadino di Paese terzo. Concludo, signor Presidente e stimatissimi colleghi, ricordando che alla Lega Nord non interessa solo rispedire a casa chi delinque o chi persiste in una condizione di illegalità: per la Lega Nord la parola d'ordine è sicurezza, non è solo quella che passa attraverso le forze di polizia, ma anche, e forse soprattutto, quella sicurezza che si può mantenere garantendo un'integrazione responsabile, basata su princìpi e su valori reali. Ecco perché ci troviamo a discutere l'attuazione effettiva e l'integrazione di tanti importanti provvedimenti, come il permesso di soggiorno a punti, la questione dei matrimoni misti e soprattutto la conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero. è il primo passo verso l'integrazione e, personalmente, ritengo che la conoscenza e il rispetto delle nostre regole sia il miglior permesso che uno straniero può dimostrare di avere sul nostro territorio. Signor Presidente, signori del Governo, quella di ieri è stata una giornata terribile sul fronte delle condizioni dei migranti e dei rifugiati nel nostro Paese; una giornata di lutto e di tragedia a Lampedusa. Se ne è parlato, e ringrazio il presidente Chiti di avere formulato parole di cordoglio, poiché c'è veramente il rischio - e dobbiamo costatarlo sempre di più - che notizie come queste trovino il Paese ormai assuefatto a tragedie simili. È ancora di ieri la notizia che in Puglia, nel Salento, c'è stato un grande sciopero, il primo in quella Regione di lavoratori agricoli immigrati contro i caporali. Caporalato è una parola antica, che ci porta alla mente le immagini in bianco e nero del cinema neorealista dell'Italia contadina e del Mezzogiorno straccione del dopoguerra, ma questa invece è una storia di oggi, di sfruttamento grave, di lavoratori vulnerabili. Ieri lo sciopero era per il rispetto della paga sindacale, che è tra i 6 e i 10 euro all'ora: questi lavoratori sfruttati lavorano giornate intere sotto il sole cocente per meno di 20 euro. Questa dello sciopero però è anche una buona notizia, perché finalmente questi lavoratori immigrati incontrano la solidarietà e la tutela delle organizzazioni sindacali. Dunque, la loro storia finalmente non sarà più solo di silenzio, di umiliazione, di sfruttamento, di illegalità, e magari forse potremo discutere con il Ministro dell'interno anche di una nuova legge sul caporalato, di permessi di soggiorno per quei lavoratori che denunciano le situazioni di illegalità e i caporali. Infine, è sempre di ieri la notizia di pesanti scontri e rivolte nel CARA di Bari: incidenti gravissimi, che hanno coinvolto le forze dell'ordine - a cui va tutta la nostra solidarietà - e immigrati africani ammassati in modo indegno nei Centri di accoglienza. Ha ragione il presidente Vendola: questi incidenti sono il frutto avvelenato della disperazione di chi, dopo lunghi viaggi della speranza, si vede invece negata proprio la speranza di un futuro per cui si è messa a rischio la vita stessa. I Centri di accoglienza, così come i CIE, in tutta Italia stanno scoppiando per l'affollamento, per i tempi interminabili della costrizione, per il limbo d'incertezza assoluta in cui si viene ad essere collocati, e per questo rischiano di determinare ovunque una moltiplicazione delle rivolte. Altro che sicurezza, senatore Mura, se questo è l'obiettivo delle vostre proposte! Si raggiunge, infatti, in queste condizioni un livello di esasperazione assoluta che deriva dal fatto, tra l'altro, che non si riesce ad ottenere un'interlocuzione minima, affidabile, con le istituzioni del Governo italiano. Il Governo in tutte queste circostanze, a Bari, a Lampedusa, continua a dimostrarsi effettivamente al di sotto delle necessità di gestione della situazione: un'incapacità che paghiamo a duro prezzo sia sul fronte della nostra credibilità nella comunità internazionale, sia anche all'interno, in quest'Italia che sta veramente male, che la Lega continua ad inondare di messaggi fondati sull'egoismo e sull'idea della tolleranza zero, messaggi privi di qualunque umanità,

Per questo, ci opponiamo decisamente a questo vostro decreto, che è stato confezionato frettolosamente e, evidentemente, sulla base di un manifesto di pura propaganda, senza alcun interesse per i problemi Non interverrò nel merito del decreto, perché lo hanno fatto gli altri colleghi del Partito Democratico. Il punto più scandaloso e drammatico resta quello del limite massimo di durata della misura di trattenimento da 6 a 18 mesi che, secondo la direttiva, non sarebbe assolutamente obbligatorio. Allora io chiedo: chi è che ha obbligato il Governo ad introdurre un periodo di 18 mesi? Perché 18 mesi per le identificazioni? Le norme di restrizione coatta per l'identificazione dei cittadini istituiscono, di fatto, la legittimazione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie: la galera per gli innocenti. È un fatto di enorme gravità e di inciviltà giuridica, che non può passare sotto silenzio. Proprio in questo Senato dove, su proposta dei radicali, per iniziativa del presidente Schifani, alla presenza del presidente Napolitano, si è svolto un convegno importantissimo sulla catastrofe umanitaria rappresentata dalle nostre carceri, noi non possiamo commettere questa ulteriore violenza ai principi costituzionali, ai principi di civiltà giuridica, nel Paese del grande e bistrattato Beccaria. Le persone rinchiuse nei CIE sono detenute senza aver commesso alcun reato. La loro colpa esclusiva è solo quella di non possedere un documento di riconoscimento legale. C'è qualcosa di profondo: come siamo arrivati a tanta aberrazione e perché? C'è qualcosa che non va, e l'indifferenza della pubblica opinione non assolve la classe dirigente di questo Paese: e, quando dico «classe dirigente», parlo certamente di noi, la tanto bistrattata casta di cui si discute.

alla classe dirigente, appunto, in senso lato. Io sono intervenuta tante volte, signor Presidente, per denunciare le incredibili vicende di violazione e vessazione a danno di giovani tunisini che si sono consumate nel CIE di Santa Maria Capua Vetere. In quel CIE, come in tutti gli altri, ha trionfato e imperversato la disumanità organizzata dello Stato e di un modello che è un *lager* a tutti gli effetti. Questi CIE si devono chiudere ovunque: bisogna cercare altre soluzioni. Non dobbiamo più chiudere migliaia di persone dietro il filo spinato, nell'impossibilità di utilizzare anche i servizi. Nonostante il Governo non sia mai venuto in Aula a rispondere alle nostre interrogazioni, nonostante si sia tentato di impedire ai parlamentari di entrare nei CIE attraverso circolari allucinanti, nonostante s'impedisca ai giornalisti di documentare quello che accade nei CIE, a Santa Maria siamo entrati, abbiamo informato, c'è stata la visita ispettiva della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato e, seppure al prezzo durissimo di una rivolta, di fatti gravissimi, del ferimento di un grande numero di persone, di una lunga detenzione in condizioni veramente disumane, il campo è stato sottoposto a sequestro dalle autorità il CIE è stato chiuso e, alla fine di un lungo percorso di assistenza legale, che si è concentrato sull'*iter* della richiesta di protezione internazionale da parte dei tunisini, tutti hanno ricevuto la sospensiva dal tribunale di Napoli e, successivamente, un titolo di soggiorno temporaneo. di soggiorno temporaneo. Questa vicenda dimostra l'assoluta incongruenza di tutte le iniziative del Governo in questo campo. Signor Presidente, tanti sono i temi su cui si potrebbe lavorare, e se e quando il ministro Maroni deciderà di farlo, troverà, a differenza di oggi, una opposizione dialogante e propositiva.

*(PD)*. Signor Presidente, signor Ministro dell'interno, colleghi, da questa discussione non può essere rimossa la drammatica realtà che le cronache di questi giorni propongono. I 25 morti nella stiva del barcone tratto in salvo la notte scorsa dalla Guardia costiera al largo di Lampedusa ci obbligano a ricordare le migliaia e migliaia di vittime delle traversate del Mediterraneo. Su questa tragica contabilità c'è incertezza, ma tutte le stime parlano di una quantità spaventosa di morti. L'UNHCR ha stimato in oltre 1.500 le persone annegate nel Mediterraneo dalla fine di marzo. Altri stimano che circa sette persone sulle 100 che salgono sui barconi dall'altra parte del Mediterraneo non arrivino vive sulle nostre coste. Si tratta di un'emergenza umanitaria forse più grave di quella che ha portato la comunità internazionale a decidere l'intervento militare in Libia. Non è possibile rimuovere questo problema e non cercare, insieme all'Europa, una risposta efficace. Non è sufficiente, come i fatti dimostrano, il soccorso in mare che Guardia costiera, Polizia e Guardia di finanza effettuano. È necessaria un'azione preventiva, che è possibile solo se si rinuncia all'idea, assurda e totalmente irrealistica, di poter bloccare le partenze. È necessario anticipare nei punti di partenza la possibilità di richiesta di asilo e offrire la possibilità di viaggi regolari e sicuri. Solo così si può fermare o almeno limitare la strage in corso. E solo così si possono combattere sul serio, e non solo a parole, i trafficanti di esseri umani. Noi chiediamo, signor Ministro, una iniziativa politica dell'Italia in questa direzione. Ma questi fatti drammatici impongono anche un'altra considerazione. Essi dicono a chi non sia completamente sordo che non si possono considerare queste persone come «migranti economici». Quando una persona affronta dei rischi così grandi, mette in gioco la propria vita affronta una probabilità cosi alta di morire, non lo fa solo per ragioni economiche. Vuol dire che è obbligato a fuggire da una situazione che considera ancora peggiore, carica di rischi ancora più gravi. E io mi chiedo se la distinzione tradizionale tra quanti hanno diritto alla protezione umanitaria e migranti economici non debba essere in queste circostanze interpretata con umanità, alla luce di quello che stiamo vedendo. Se non affronteremo questo problema mettiamo pure in conto la moltiplicazione delle proteste, delle rivolte, e della stessa violenza che spesso le caratterizza, come abbiamo visto ieri a Bari e a Crotone, ma che si era già manifestata, e in forme non meno gravi, pochi giorni fa in un Centro considerato modello come quello di Mineo, in provincia di Catania. Le scelte che il Governo, e in particolare il Ministro dell'interno, hanno compiuto per gestire il fenomeno degli arrivi dal Nord Africa, si sono dimostrate sbagliate. La concentrazione in pochi Centri di migliaia di persone ha inceppato il funzionamento delle commissioni territoriali, che in passato avevano funzionato discretamente e che non sono state potenziate come era necessario. Gli indirizzi sempre più restrittivi nella concessione dell'asilo o di altre forme di protezione umanitaria hanno fatto il resto. Noi chiediamo al Governo che, se non intende ascoltare gli argomenti della solidarietà, ascolti almeno quelli del realismo e corregga un indirizzo che è destinato a produrre nuove sofferenze e nuove tensioni. D'altronde, l'esperienza dovrebbe pur dirvi qualcosa se è vero che oggi in qualche modo, con questo decreto, siete obbligati a ritornare su decisioni che si sono dimostrate fallimentari. voglio dire l'ultima cosa, signor Ministro e cari colleghi, sul prolungamento a 18 mesi del trattenimento nei CIE. Vi ripeto una cosa già detta: andate una volta a vedere con i vostri occhi di cosa stiamo parlando. Ministro Maroni, una volta metta piede e vada a vedere con i suoi occhi in quei CIE, dove lei non è mai entrato durante tutti questi anni! Il prolungamento della detenzione è una misura costosa e totalmente inefficace. Tutti i dati disponibili dicono che il numero di effettive espulsioni cala con il crescere del tempo di trattenimento e che esse sono percentualmente diminuite in misura significativa già con il passaggio da 60 a 180 giorni. Ma non ci sono solo ragioni di efficacia, bensì anche di principio. Uno strumento che poteva servire per favorire l'allontanamento dall'Italia di responsabili di gravi reati lo avete fatto diventare un modo per tenere prigioniere persone che non hanno commesso altro reato che il tentativo di fuggire dalla miseria. Nei CIE avete messo nelle stesse stanze condannati per reati gravi e ragazzini incensurati, appena maggiorenni, e si tratta di una struttura che viola diritti umani fondamentali. Ho detto, e ripeto, che i CIE sono peggiori del peggiore dei anche nel peggiore dei penitenziari, fino a quando la Costituzione italiana resterà in vigore, lo Stato, almeno in linea di principio, non può limitarsi a recludere e custodire una persona;

non è solo un numero. Per i reclusi nei CIE, invece, non c'è niente di tutto questo: sono tenuti in gabbia e basta, il loro è un tempo vuoto, una parte della vita semplicemente rubata e il loro essere persone viene negato. settimane, ma di 18 mesi, si tratta di una parte importante della vita di una persona: il fatto che pensiate di tenere per 18 mesi migliaia di giovani uomini e giovani donne nelle stesse strutture, con la stessa organizzazione, con gli stessi servizi di quando il limite era di 60 giorni, dice da solo della vostra assoluta indifferenza alla questione dei diritti delle persone. E questo accrescerà, non risolverà i problemi. Sono queste alcune

sono il frutto avvelenato della disperazione di chi, dopo lunghi viaggi della speranza in fuga da guerra, persecuzione e fame, si vede negata la possibilità di un futuro di accoglienza. Le insopportabili attese per le pratiche di valutazione delle richieste d'asilo e il numero crescente di dinieghi rappresentano una condizione inaccettabile

della discussione generale sul disegno di legge sui rimpatri. L'articolo 10 della nostra Carta costituzionale sancisce solennemente che «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge».

essere accolto dal nostro Paese e «ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge». In Italia c'è una legge che rispetta i diritti umani; noi non siamo la Libia che non li rispetta, noi non firmiamo i Trattati con la Libia che non rispetta i diritti umani. Noi li rispettiamo e li condividiamo, ma trattiamo quelle persone come animali. Nei CIE, dove anche il Ministro con i suoi occhi ha potuto vedere

dire all'opinione pubblica la vostra posizione, cioè che non li volete. Ed è una cosa vergognosa, questa. È vergognoso dover dire all'opinione pubblica che abbiamo un Governo che respinge

a leggere e a rispettare, cioè l'articolo 10 della nostra Carta costituzionale, perché solo così si può capire la disperazione di queste persone.

li vogliamo solo cacciare via, senza un ordine, senza un cuore. Non mi meraviglio, un Governo che ha firmato un Trattato di amicizia, lo ripeto, con la Libia, che non rispetta i diritti umani, solo questo poteva fare, è questo che contrasteremo sempre. Noi in questo mese andremo nei Centri di accoglienza, chiamiamoli così, per verificare quello che abbiamo visto e quello che anche il Ministro ha confermato di aver visto, un Centro che non è accogliente, un Centro che vuole far capire che questo Paese non intende rispettare i diritti umani, ma cacciare persone che soffrono. Noi questo non glielo permetteremo.

È «fatta di sensori e telecamere che captano ogni movimento lungo la frontiera. Popolare presso l'elettorato americano (il 68 per cento l'approva), il muro in meno di 15 anni è stato silenzioso testimone, tra il deserto di Sonora e quello dell'Arizona meridionale, di almeno 5.000 morti tra migranti: il macabro conteggio è *bipartisan*» (della Commissione nazionale dei diritti umani messicana e dell'Unione delle libertà civili americana).

foto di una recinzione di filo spinato particolarmente difficile da superare. Questo accade negli altri Paesi, mentre noi siamo alle prese con i soliti problemi, con una valutazione della sinistra di una politica dell'accoglienza indiscriminata, senza regole. Ci troviamo a dover affrontare ciclicamnte gli stessi problemi. Aggiungo, sempre per cercare di sollevare i colleghi dall'ascolto pesante di argomenti importanti, anche un altro articolo, questa volta sull'inserto «D» de "la Repubblica",

Dice Rampini, *radica-chic*: «Ho provato a immaginarmi una scena simile nella mia New York. Impossibile. Un solo viaggiatore senza biglietto che rifiuti di pagare la multa al controllore farebbe scattare reazioni poderose. La polizia arriverebbe in forze, armata fino ai denti. L'umiliazione la soffrirebbe l'abusivo. Che non finirebbe il viaggio su quel treno, e sarebbe in manette prima di arrivare a destinazione

parte della politica italiana che continua ad assumere questi atteggiamenti: da un lato, chiede l'arresto di un immigrato che va su un treno senza biglietto, sostenendo che un tale comportamento negli Stati Uniti sarebbe poderosamente e rigorosamente

ha valutato negativamente dal punto di vista politico il lavoro che avevamo fatto con grande attenzione nel 2008 e nel 2009: ha ritenuto cioè che quel pacchetto sicurezza 2008-2009 avesse raggiunto i suoi obiettivi di effettività delle procedure di espulsione, stava dando dei risultati importanti in termini di numeri. E allora quella corrente ideologico-politica ha iniziato a ragionare su come smantellare quel lavoro. stamattina un giornalista ci chiedeva se fosse un complotto. Io ho risposto di no, perché i complotti avvengono all'ombra, senza essere scritti da nessuna parte. se voi frequentate alcuni siti *web* (ce n'è uno in particolare che si chiama «www.penalecontemporaneo.it», troverete a partire da ottobre del 2010, quindi ben prima della scadenza del termine di attuazione della direttiva rimpatri, un'analisi di questa corrente politico-ideologica che sostanzialmente dice che deve smantellare l'apparato sanzionatorio repressivo messo in campo per procedere all'espulsione degli stranieri. E dove arrivarci utilizzando tutti i percorsi possibili. E così hanno fatto, passo dopo passo. Sono riusciti dapprima a convincere alcune procure, che hanno iniziato a cogliere l'opportunità della scadenza dei termini di attuazione della direttiva rimpatri per ritenere che quelle fattispecie incriminatrici della inosservanza dell'ordine di allontanamento, che avevano funzionato, dovevano essere disapplicate. siamo rimasti davvero basiti a vedere che delle procure della Repubblica che sono chiamate ad applicare la legge, addirittura promuovano circolari dirette a farla disapplicare dai propri procuratori *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL)*, addirittura invitando, anche in maniera forte, le forze dell'ordine a non convalidare più gli arresti. Questo, nonostante ci fosse una minoritaria dottrina, sempre in quel sito (andate a vedere: c'è un unico magistrato che ha avuto il coraggio di dirlo. Si chiama Tomaso Epidendio; lo dico qua perché rimanga agli atti che un magistrato serio, che ha cercato di dire ai propri colleghi che forse stavano esagerando, c'è) che rilevava come la direttiva rilevava come la direttiva rimpatri fosse stata adottata prima del Trattato di Lisbona, e che dunque non poteva in nessun modo incidere sulla potestà sanzionatoria penale dello Stato, e dunque non poteva entrare nella materia penale, può riguardare l'aspetto delle procedure amministrative, ma non quello delle fattispecie incriminatrici. Leggetevi questi articoli di Tomaso Epidendio, che cerca di dire ai propri colleghi: ragazzi, cerchiamo di darci una controllata, perché stiamo davvero esagerando; stiamo andando al di là del compito che ci dà la Costituzione: che è di perseguire i reati, e non di capovolgere la volontà popolare democraticamente

da un collegio con un giudice italiano (Antonio Tizzano, professore di diritto comunitario) che non ha mai amato le politiche che iniziavamo ad applicare in questo Stato, è stata colta l'occasione per fare una sentenza dove ovviamente il tema la Corte di giustizia sorvola su questo aspetto, forse avrebbe dovuto dedicarvi qualche riga in più invece che una riga sola. ma il diritto comunitario prevale sul diritto interno, e quindi la direttiva rimpatri porta alla disapplicazione, disapplicazione, anzi all'abrogazione delle fattispecie incriminatrici. Ho qui una trentina di sentenze che scientificamente hanno riguardato tutti gli aspetti che stavano funzionando, da ultimo quello, citato, del matrimonio del clandestino. Abbiamo detto che lo *status* di clandestinità è un reato, così come accade in tutti Paesi europei e l'abbiamo già dimostrato. La Francia, che ha attuato la direttiva rimpatri, non ha modificato di una virgola il reato di clandestinità, per il quale si prevede addirittura l'arresto fino a un anno, oltre che l'ammenda. Ebbene, noi in sostanza abbiamo stabilito che un clandestino, proprio perché sta commettendo un reato, non può presentarsi davanti a un ufficiale di stato civile e chiedere la pubblicazione degli atti di matrimonio. Appare davvero qualcosa

di sentenze che scientificamente e con motivazioni di stampo prettamente politico hanno cercato, e in parte ci sono riuscite, di smantellare questo pacchetto sicurezza. Con il decreto-legge in esame cerchiamo di riproporre queste posizioni,

continuiamo nella nostra politica di repressione dell'immigrazione irregolare. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo nella discussione sulla conversione in legge di questo decreto con animo turbato per quanto avviene nella mia Regione, la Puglia. Non mi riferisco solo agli scontri di Bari, dove una situazione insostenibile ed inconcepibile ha dato i risultati che sappiamo in termini di ordine pubblico e di danni alle cose e alle persone, ma anche a quello che succede a Nardò, dove i lavoratori agricoli extracomunitari sono in sciopero per il rispetto dei loro diritti. Si tratta di vicende diverse e controverse, che nella loro complessità spiegano quanto sia inadeguata e nociva la rozza semplificazione del Governo, di cui questo decreto è esemplare articolazione. Da anni la destra ha in materia di migrazione e di migranti una posizione demagogica e miope, tesa a sfruttare le ansie di un'opinione pubblica impaurita. Ma più di un decennio di ossessione securitaria, di proclami criptorazzisti, di decreti e di leggi speciali...

Senatore Gramazio, la richiamo all'ordine per la seconda volta.

fortemente discutibili, sia dal punto di vista del diritto internazionale e costituzionale, sia da quello del diritto naturale, non ha in alcun modo migliorato la situazione, e i fatti di Bari e di Crotone di ieri lo dimostrano. Fra i grandi Paesi europei, l'Italia è quello che ha il numero relativamente più basso di immigrati, ma anche quello dove si verificano le maggiori difficoltà di convivenza. Anche in questo decreto si fa fatica ad individuare non dico una strategia, ma un abbozzo di politica, un nocciolo di idee. Come tutti gli scolari che non hanno studiato, il Governo prende tempo, mena il can per l'aia, si arrampica sugli specchi. Ha forse un altro l'allungamento a 18 mesi del termine per esaminare le richieste di asilo? Può essere definita in altro modo l'irrogazione di una pena detentiva senza processo e senza delitto? Con questa alzata di ingegno il nostro Governo ritiene di potersi esimere dagli obblighi contenuti nelle dichiarazioni, nelle Convenzioni e nei Trattati internazionali cui abbiamo aderito. In questo, come dicevo, c'è un'esemplare coerenza rispetto all'azione complessiva di questo Dicastero presieduto dall'onorevole Berlusconi, ammesso che lo presieda ancora e non abbia già passato il testimone all'onorevole Maroni o ad altri. Questo Governo, onorevoli colleghi, ha l'abitudine dell'annuncio e quella parallela della rimozione: promette ciò che non farà e nasconde ciò che effettivamente fa. Per il Governo, per il Ministro dell'interno, basta che non si sappia in giro: diversamente, perché proibire l'ingresso nei CIE e nei CARA dei giornalisti, con un rigore che non viene applicato nemmeno nelle carceri? Perché è ferma convinzione dei nostri governanti che un problema esiste solo se compare in televisione; quindi, via le telecamere, via la questione. Magari fosse così, magari bastasse questo, onorevoli colleghi. Abbiamo bisogno di altro, di nuove e meno sgangherate idee per fare i conti con temi epocali. repressiva, che è certo necessaria in alcune situazioni, finisce, se lasciata da sola, per moltiplicare ed aggravare i problemi. Non è facendo il «gioco delle tre carte» con i disperati che fuggono dalla guerra e dalla fame che renderemo più sicure le nostre città e i nostri territori; non è nascondendo la polvere sotto il tappeto che renderemo la nostra casa più pulita; lo faremo ampliando l'area della visibilità e della protezione sociale, mettendo le istituzioni al fianco dei lavoratori agricoli stranieri in lotta nel Salento; lo faremo, caro ministro Maroni, modificando il decreto flussi, che è quasi inapplicabile. Voglio ricordare ai colleghi che questo è il mese della raccolta del pomodoro: ci sono migliaia di migranti sulle nostre terre e certamente non sono arrivati per il decreto flussi. Tutte le aziende agricole che hanno fatto richiesta quattro mesi fa stanno ancora aspettando questi lavoratori. Mi chiedo quale sia il meccanismo più agile, facile e agevole per far incontrare la domanda e l'offerta e lo chiedo al ministro Maroni, che insiste sempre

per coloro che assumono gli schiavi. Ci abbiamo provato nella precedente legislatura: il disegno di legge fu approvato dal Senato ma la caduta del Governo rese impossibile portare a casa questo provvedimento, che abbiamo pertanto ripresentato qui al Senato voglio ringraziare tutti coloro che lo hanno sottoscritto, senatori che appartengono a più forze politiche). Concludo in due parole, signor Presidente: voteremo con convinzione contro la conversione di questo decreto. Penso che anche tale provvedimento dimostri dimostri che un Centro di identificazione ed espulsione, politicamente parlando, dovrebbe occuparsi al più presto di questo Esecutivo, senza documenti e, ahimè, senza idee. *(Applausi

in quanto mi si offre la suggestiva opportunità o occasione di assistere alla trasposizone in legge nazionale di una direttiva, la n. 38, di cui fui relatore davanti al Parlamento europeo. Considero quindi questo momento una sorta di esame, tardivo, dopo sette anni, ma quantomeno opportuno, della validità, dello spirito, delle idee e soprattutto del voto di quelle giornate davvero tumultuose. Il dibattito durò infatti un anno e riuscimmo ad approvare questa direttiva solo un mese e mezzo prima della scadenza della legislatura; di allora, di 15 Paesi e circa 650 parlamentari, fosse difficile immaginare di ottenere un consenso unanime. Eppure, dopo sette anni, scopro con piacere che le idee di allora sono ancora

signor Ministro, temutissima da tutta Europa, tant'è che la Commissione europea inventò un modo per controllare nei primi tre mesi di apertura il via vai di questi immigrati. Si temeva un esodo biblico dei cittadini dai 12 Paesi PECO,

anziché andare loro in Europa, era l'Europa che entrava a casa loro, con una somma di incentivi e di aiuti che a quel punto avrebbero consentito loro di rimanere profittevolmente in Patria con grandi prospettive. Questa direttiva fu aiutata da queste considerazioni, altrimenti l'apertura che proponeva avrebbe rappresentato davvero un momento di grande problematicità.

in questa sede si parli anche della direttiva 2008/115, che regola le ipotesi di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi in situazioni irregolari. Molte idee sono state perfezionate

i principi di un'umana partecipazione al dramma delle persone che ne sono interessate. Cominciamo dal permesso di soggiorno. La direttiva - questo è un aspetto forse poco considerato

poi un altro concetto che fu introdotto, non senza scossoni, nel dibattito, vale a dire la necessità di garantire risorse economiche sufficienti per ottenere il permesso di soggiorno. previsione fu interpretata da alcuni come una limitazione della libertà condivisa da tutti, e quindi come una selezione, una discriminazione. il passare del tempo si ebbe però l'occasione di verificare appieno l'opportunità di questa misura, proprio per garantire la serietà del provvedimento e la certezza del diritto. Non dimentichiamo che quando parliamo di permesso

Anche in questo campo, signor relatore, la direttiva n. 38 ebbe un coraggio che in altri tempi non sarebbe stato nemmeno immaginabile: dimezzò i tempi per la cittadinanza

con una certificazione, che da un Paese terzo raggiunge il cittadino comunitario. Questa è stata un'apertura davvero importante e ho visto la precisazione che viene fatta nel che rispecchia il principio e lo spirito della direttiva: lo precisa meglio quando parla di relazione stabile ufficialmente attestata, per quanto riguarda la documentazione e la dimostrazione del rapporto familiare che è derivante da una situazione di convivenza o dipendenza per vari motivi, a volte anche per motivi di salute ed economici e motivi di studio

della sorveglianza: qui si parla di verifica delle condizioni di soggiorno solo per l'insorgenza di ragionevoli dubbi o di eventi che possono disturbare l'ordine pubblico.

furono introdotti condizionamenti ben più garantisti rispetto a quelli precedenti, proprio per quanto riguarda il criterio dell'espulsione di qualche immigrato qualche immigrato resosi colpevole dei fatti previsti dalla normativa, e anche ripresi dal provvedimento nazionale: reati gravi e appartenenza ad associazioni mafiose, a organizzazioni terroristiche, a partiti messi all'indice, oppure a qualcosa che crei pericolo per la

che questo passaggio, nella direttiva n. 38, ha una radice italiana. I primi a fare il tifo per un maggior garantismo nei casi di espulsione furono gli immigrati italiani nel Nord-Europa, che si fecero vivi durante il dibattito. Si erano verificati alcuni casi di facili espulsioni di immigrati - guarda caso - italiani, in particolare nelle Regioni Nord-occidentali della Germania, dove, per un banale furto, venivano espulsi figli e nipoti di immigrati nati e residenti da sempre in Germania. In quel caso c'era evidentemente un accanimento, che veniva interpretato come tale da organizzazioni di emigrati. Introducemmo pertanto questo principio di cautela, sia nell'identificazione delle cause di eventuale espulsione, concedendo a chi viene colpito da provvedimento di espulsione dalle autorità di un Paese membro la possibilità di ricorrere alla Corte di giustizia di Lussemburgo che ha l'ultima parola, soprattutto su casi che che possano interessare la sicurezza dello Stato. Solo in questi casi la Corte potrebbe o potrà approvare un provvedimento di espulsione: credo che ciò sia un passo avanti notevole per chi vuole la certezza del diritto fino in fondo. Di qui, poi, il passaggio

Qui ci sono molti colleghi, anche dell'opposizione, con cui dividiamo l'esperienza al Consiglio d'Europa, dove ad ogni assemblea e sessione si parla di queste problematiche con sempre maggiore insistenza e con sempre minore informazione corretta. Questa è la ragione per cui ho proposto - il Ministro lo sa perché mi ha aiutato in questo, assieme alla collega Maraventano - una delegazione del Consiglio d'Europa, con cui siamo andati a Lampedusa e abbiamo visitato i Centri di accoglienza: abbiamo vissuto per due giorni e mezzo l'attività

vengono accolti gli emigrati provenienti da zone sub-sahariane, quelli colpiti dal pericolo reale di guerra civile o comunque di incolumità personale. Vengono rimandati a casa solo i cosiddetti emigrati economici, protagonisti di un tentativo di emigrazione che serve a migliorare le condizioni della vita, ma che non fuggono da un pericolo per la loro vita stessa. Quindi, già a Lampedusa c'è questo primo coraggioso *screening*, ma è chiaro che tutto questo richiede anche un certo tempo. C'è un controllo concreto, fisico, con strumentazioni all'avanguardia, elettroniche, ma comunque è sempre un'operazione molto delicata. Ecco perché la polemica sui 18 mesi non mi coinvolge più di tanto: considero i 18 mesi un tempo limite, ma vorrei segnalare ai colleghi

ormai consolidato, e vedo che questa legge ne è la prova. L'applicazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione - che dobbiamo cercare di gestire bene - è un passo avanti importante per tutta la problematica che riguarda le espulsioni. Vorrei anche ricordare,

titolari di un diritto di libera circolazione; abbiamo dato i soldi per il viaggio, i soldi per un'autonomia quotidiana. Peccato che siano stati fermati alle frontiere, in particolare quelli che volevano andare in Francia, vale a dire oltre il 50 per cento degli emigrati. Per questo davvero approfondire il dialogo con l'Europa, non solo attraverso il Consiglio d'Europa, ma attraverso la Commissione europea. Aggiungo che, con il Consiglio d'Europa, la settimana scorsa siamo stati nei campi profughi della Turchia, dove stanno confluendo a migliaia i profughi della Siria. il dramma di oggi, il sangue che scorre nelle strade siriane si riverserà ancora di più sulla Turchia. Dunque è un problema anche di altri Paesi. Va detto che la Turchia non riconosce lo *status* di rifugiato, in quanto non ha firmato certi capitoli del Trattato di Ginevra del 1951; però la Turchia oggi è ammirevole per impegno concreto, per spiegamento di forze e per spirito di solidarietà nell'accoglienza. Oggi i profughi sono 10.000, in sette campi diversi,

una lagnanza diffusa sul fatto che c'è una notevole indifferenza da parte di certi Stati. Signor relatore, quale sorpresa? Già al momento del varo di queste direttive, Danimarca, Olanda e Svezia posero l'*opting out*, vale a dire l'opzione del va bene ma noi non ci stiamo, su questa materia applichiamo le nostre leggi nazionali; abbiamo regole nostre, e quelle che decidete come Comunità non ci appartengono, o le prendiamo dove possiamo. Questi Paesi oggi devono essere coinvolti, non solo sul piano del diritto o della richiesta di aiuti finanziari ed economici per i profughi, ma della politica pura. È una decisione politica che devono prendere, e devono prendersi parimenti le quote di immigrati che spettano loro: soprattutto Paesi come Francia, Germania e Regno Unito, dove vuole andare la stragrande maggioranza di coloro che approdano a Lampedusa. concludere, senza permettermi di interferire o commentare l'aspetto giuridico (che il nostro relatore ha interpretato in maniera corretta, esemplare e coerente, con bellissime indicazioni politiche), richiamando lo spirito di queste direttive, che si rispecchia, con i correttivi che ho cercato di ricordare, con quello che oggi stiamo vivendo anche in questa Assemblea. Lo spirito che dobbiamo trasmettere trasmettere agli altri Paesi europei è quello della solidarietà, dell'accoglienza, dell'integrazione, dello spirito di umanità fino al massimo livello, ma con tutte le attenzioni e le prudenze del caso.

non faremmo che far trasferire questi poveretti da un'emergenza ad un'altra, poco conta se condivisa con noi. L'Europa si sta impegnando solo sul piano finanziario;

di vivere queste giornate; sono eroici i suoi abitanti, e lo sono tutti coloro che si stanno occupando dell'accoglienza e dell'emergenza. Per questo, desidero chiedere al Presidente di aggiungere la mia

parere non ostativo». « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, prendendo atto dei chiarimenti forniti dalla Ragioneria generale circa la correttezza contabile della copertura di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, in quanto predisposta su risorse in conto residui di stanziamento, peraltro rinvenienti da una preesistente autorizzazione di spesa e riversate su apposita contabilità speciale nel corso del 2011, già scontati sugli effetti stimati sui tendenziali a legislazione vigente. Osserva tuttavia che tale copertura si prefigura come non perfettamente conforme alle modalità previste dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 3.2 (limitatamente al comma 3.4, 3.18, 3.51, 3.100, 3.48, 3.101 (testo 2) e 3.103. Esprime altresì parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.2-a. 3.6, 3.17, 3.0.1 e 3.102. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti».

Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha apportato modifiche al calendario corrente con l'inserimento all'ordine del giorno, per domani, alle ore 17,30, di un'informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sulla situazione economica. Dopo l'intervento del Presidente del Consiglio, i Gruppi potranno intervenire per dieci minuti ciascuno. È stato chiesto alla RAI di provvedere alla trasmissione di un riassunto dei lavori.

Domani mattina si passerà all'esame degli ordini del giorno e alle votazioni finali del rendiconto e del bilancio interno. Seguirà, sempre in mattinata, l'esame degli altri argomenti già previsti dal calendario, modifica allo statuto del Fondo monetario internazionale. È stata infine richiesta al Governo la disponibilità a rendere un'informativa sulla situazione in Siria.

mentre, per quanto riguarda i dispositivi, vi sono alcune proposte di riformulazione. Iniziando dall'ordine del giorno G100,

secondo capoverso nella seguente maniera: «ad attivarsi celermente per migliorare sempre più le condizioni dei migranti presenti nei Centri di identificazione ed espulsione, nei Centri di accoglienza nonché nei Centri accoglienza dei richiedenti asilo, consentendo, finita l'emergenza, l'accesso anche ai giornalisti ne propone la seguente riformulazione: «a rendere accessibili, ai sensi della legge n. 241 del 1990, gli atti relativi alla gestione dei Centri al fine di consentire una migliore informazione sull'amministrazione e la gestione delle strutture in questione».

ovviamente sempre considerando finita l'emergenza: «si impegna il Governo a: predisporre ed adottare tutte le misure necessarie a consentire ai giornalisti e agli operatori dell'informazione l'accesso ai centri per immigrati e richiedenti asilo, modificando le regole d'accesso».

G104, il parere è contrario sulle premesse, mentre è favorevole sul dispositivo, senza modifiche.

*(PD)*. È un po' paradossale che mi si chieda di togliere proprio la parte che prevede la presentazione (e quindi il coinvolgimento del Parlamento) di una relazione

ricordare al Governo, che ha chiesto solo una minima riformulazione, che cosa chiede l'ordine del giorno G105: esso impegna il Governo «ad esigere in tutte le competenti sedi internazionali, a partire dal Consiglio dell'Atlantico del Nord,

sia una questione interna di partito, ancora prima che di maggioranza, però occorre mantenere un minimo di decenza. Vi siete impegnati «ad esigere». Voglio proprio vedere come farete ad esigere.

VIALE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei ricordare che il Ministro, con nota dell'8 aprile 2011, ha comunque ribadito l'accesso ai Centri per immigrati presenti su tutto il territorio nazionale ai parlamentari europei, ai deputati e ai senatori della Repubblica.

il Ministro, con circolare dell'8 aprile 2011, lo ha già ribadito. Cosa diversa è per quanto riguarda i giornalisti,

un'ultima precisazione (può essere banale, ma per noi non è tale): la frase «finita l'emergenza» cosa vuol dire per voi? Quand'è finita l'emergenza? A rigore e normativamente, c'è uno stato di emergenza dichiarata con un provvedimento *ad hoc*, a cui ci si può richiamare, finita l'emergenza, così come dichiarata. Colleghi, il Parlamento esiste per questa forma di confronto. È un dibattito.

Presidente, intervengo sull'ordine del giorno G105, esprimendo l'auspicio e l'augurio che il Governo non voglia accoglierlo, essendo di

Ci meravigliamo che il Governo possa aver espresso parere favorevole in presenza di molte dichiarazioni, anche in sedi formali come le Commissioni e l'Aula della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da parte dei Ministri della difesa e degli affari esteri che, di fronte a richieste di questo tipo, hanno sempre espresso l'assoluta contrarietà del Governo, anche per le ragioni evidenti di rapporto con i nostri alleati. Un'alleanza come la NATO non ha alcuna competenza e non può, in alcun modo, essere impiegata in chiave di prevenzione

Le forze navali schierate davanti alla Libia devono servire a prevenire l'ingresso illegale di armi in Libia, in violazione delle norme sull'*embargo* di fornitura di armi al regime di Gheddafi. Non hanno evidentemente alcuna possibilità pratica, oltre che giuridica, di fermare i barconi dei disperati. È evidente che questo è un ordine del giorno di cattiva propaganda, signor Ministro, e ci auguriamo che l'Aula del Senato lo respinga con fermezza. Senatore Pedica, ha risolto il problema?

seguente frase: «ferma restando la possibilità di concedere specifici permessi, anche in condizioni di emergenza, ai giornalisti»,

l'interno*. Confermo la proposta di riformulazione. Vorrei ricordare che comunque

Save the children, della CARITAS, nonché tutte le associazioni che hanno in corso con il Ministero dell'interno progetti in fase di realizzazione nelle strutture di accoglienza finanziati con i fondi nazionali ed europei. Noi riteniamo che la presenza dei giornalisti sia un fatto importante di comunicazione e di libertà. anche *una tantum*, la possibilità di intervenire come informazione, la cosa ci fa preoccupare molto, perché, oltre a tutte le organizzazioni, c'è anche la possibilità di avere la libertà di far vedere qualcosa. Ciò ci ci crea il dubbio di non volere informare l'esterno, se non attraverso organi che non hanno uno strumento che può rendere visibile ciò che alcuni occhi vedono. È un

Metto ai voti l'ordine del giorno G100,